colleghi, il sottosegretario Mantica, intervenendo lo scorso luglio nella III Commissione affari esteri della Camera nel dibattito sulla risoluzione presentata dall'onorevole Franco concernente il processo di razionalizzazione della rete consolare italiana, faceva presente la disponibilità del Governo ad un dialogo costruttivo con il Parlamento su un tema così delicato e significativo per la proiezione internazionale del nostro Paese. A ben vedere, questo è lo scopo fondamentale della mozione illustrata ieri dal senatore Micheloni: mantenere forte e costante un dialogo tra Parlamento ed Esecutivo, dal momento che sono in gioco questioni di particolare rilevanza sia per quanto riguarda le relazioni con i residenti italiani all'estero, sia per tutto ciò che attiene a rapporti commerciali, culturali ed economici di primo piano per l'Italia. In buona sostanza, si ribadisce la necessità che il Parlamento sia chiamato in prima persona a valutare e discutere il piano di razionalizzazione della nostra rete diplomatica e consolare anche a supporto delle gravose decisioni che, indubbiamente, il Governo è chiamato ad assumere. Da questo punto di vista, non posso fare a meno di rilevare che, alle prime notizie concernenti il citato piano di ristrutturazione - notizie risalenti alla metà del corrente anno, cui hanno fatto seguito numerose proteste e rimostranze da parte di vari organismi e dopo l'approvazione di una specifica risoluzione alla Camera dei deputati, nulla si è modificato - a mio giudizio - nell'atteggiamento politico del Governo. Infatti, a quanto è dato sapere, recentemente quella prima definizione del piano avrebbe subito delle modifiche volte a sostituire alcune sedi consolari soggette a possibile chiusura con altre, mantenendo comunque inalterato il risultato finale, con ciò confermando l'impostazione iniziale tesa a produrre una serie di soppressioni di sedi senza alcuna possibile e condivisa valutazione delle eventuali incidenze negative, soprattutto con riferimento alla presenza di nostri connazionali in quelle realtà, e delle possibili ripercussioni nei rapporti politici, economici e culturali tra l'Italia e i Paesi interessati dalle chiusure. Come è noto e come dimostrano alcune manifestazioni di protesta in corso in queste ore in Svizzera e in altri Paesi, anche la "seconda" (uso la parola seconda tra virgolette) versione del piano del piano di razionalizzazione sta provocando diffuso malcontento tra i nostri connazionali interessati dal provvedimento, così come tra quelle realtà economiche e culturali che hanno rapporti consolidati con il nostro Paese. Si dà il caso, ad esempio, che in Germania il presidente del Saarland, come già ricordato in sede di illustrazione del documento al nostro esame, si sarebbe perfino reso disponibile ad offrire gratuitamente l'uso di alcuni locali di proprietà dell'amministrazione per mantenere in attività in quella regione una struttura di servizio per i nostri connazionali residenti. Si propone perciò, signor Sottosegretario, all'attenzione del Parlamento e del Governo la necessità che il piano di razionalizzazione consolare corrisponda ad alcuni precisi criteri Detto piano non può essere unica prerogativa degli uffici direzionali del Ministero. Esso deve realizzarsi con un reale processo condiviso tra tutte le istituzioni coinvolte e, certamente, con il primario obiettivo di consolidare una marcata presenza del nostro Paese nei nuovi mercati mondiali, tenuto conto, in particolare, anche del nostro turismo e delle nostre attività commerciali. Deve però, e non da ultimo, garantire i necessari servizi alle comunità italiane residenti all'estero, anche utilizzando tutte le possibili innovazioni tecnologiche per rendere più efficaci ed efficienti tali servizi. Da questo punto di vista credo si tratti di operare con la consapevolezza che il processo di razionalizzazione degli uffici consolari non può trasformarsi in un semplice atto amministrativo. In questo quadro è del tutto evidente che la rete dei consolati deve rispondere anche al criterio della presenza dei cittadini italiani nel mondo. Allo stesso tempo va garantito ogni servizio, anche per il tramite di agenzie consolari o di uffici presso le autorità locali, a quei nostri connazionali che dovessero trovarsi in una situazione di difficoltà per la chiusura di uffici vicini alla loro residenza, così come va dato ulteriore stimolo al processo di informatizzazione delle strutture consolari al fine di prestare servizi efficienti in tempi ragionevoli. Concludendo, signor Presidente, questa è l'ispirazione che muove la nostra parte politica su un tema che sta suscitando molta preoccupazione fuori dai nostri confini, fra le comunità e gli stessi Paesi dove da sempre è viva la presenza dell'Italia. Sono convinto però che esistano tutte le condizioni per una comune iniziativa volta a garantire le prerogative parlamentari e la stessa autonomia decisionale dell'Esecutivo, in un contesto molto spinoso e nel quale si tratta di prestare grande attenzione, certo, alla proiezione estera del nostro Paese, non dimenticando però le condizioni materiali e sociali in cui si trovano a vivere circa 5 milioni di nostri connazionali in realtà spesso fra loro

Signor Presidente, onorevole sottosegretario Mantica, onorevoli colleghi, l'Assemblea del Senato è chiamata oggi ad esprimersi su una questione di grande importanza per le nostre collettività residenti all'estero. L'Italia si appresta ad attuare, tra la fine del 2009 e il 2011, un'iniziativa governativa riferita al processo di razionalizzazione della rete degli uffici consolari all'estero. Premetto che condivido pienamente la mozione del senatore Micheloni, alla quale chiedo di aggiungere la mia firma. Per quanto riguarda il coinvolgimento del Governo all'interno del Parlamento, in merito alle modalità di razionalizzazione degli uffici diplomatico-consolari, credo sia opportuno approfondire l'argomento gradatamente e scrupolosamente. Non amo parlare di razionalizzazione, se questo termine implica un indiscriminato taglio delle risorse, ma preferirei intenderlo come una progressiva riorganizzazione del sistema. Da quanto espressamente annunciato dal sottosegretario Mantica, il processo di razionalizzazione prevede la chiusura di 13 consolati nel territorio europeo, 2 negli Stati Uniti d'America, 2 in Australia, 1 in Sudafrica, la chiusura dell'ambasciata di Lusaka in Zambia, il declassamento di 4 consolati generali a consolati (Alessandria d'Egitto, Basilea, Gedda e Karachi). Se quanto dichiarato dovesse concretamente realizzarsi, ciò significherebbe un forte insuccesso della nostra presenza all'estero e sarebbe, per noi, un duro colpo alla storia dell'emigrazione italiana. L'esistenza della rete consolare ha permesso in questi anni di svolgere un ruolo istituzionale di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le cariche diplomatico-consolari. È stato infatti possibile valorizzare il loro ruolo nei confronti sia delle collettività, sia dell'autorità consolare. Si parla di «consolato digitale», di «servizi consolari a distanza» e di rilascio «del passaporto biometrico digitale»: tutto questo sta alla base di un progetto che mira a consentire ai nostri connazionali di non spostarsi più dal proprio luogo di residenza, avendo così la possibilità di poter interagire con la pubblica amministrazione. Mi domando: come possiamo giustificare la chiusura delle reti consolari ai nostri emigrati? Come possiamo pretendere che le persone più anziane vadano su Internet per prendere un appuntamento che prima era garantito da un personale qualificato e diventato, per loro, nel tempo, un importante punto di riferimento? Esistono certamente nuove esigenze, ovvero l'avvio alla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare in considerazione del mutato contesto geopolitico. Se questa prima era di carattere politico-economico, ora si muove anche in ambito commerciale. commerciale. Fondamentale è il ruolo che svolgono le ambasciate e i consolati che, affiancandosi alle imprese con scopi collaborativi, si pongono anche come punto di riferimento per mantenere sempre vivo il contatto con la madrepatria. Il nostro Governo giudica eccessive le uscite finanziarie legate a questi rapporti, ma sicuramente la politica dei tagli non è quello di cui la struttura consolare ha bisogno. Tanto meno tutto ciò può tradursi in una riduzione dei servizi per migliaia di nostri connazionali, i quali invece hanno bisogno di sentirsi ancora parte integrante di questo nostro con cui sarebbe giusto avessero una continuità di dialogo. Ed è in questa occasione che sollecito il Governo ad avviare quanto prima un dialogo con le Commissioni parlamentari competenti, al fine di adottare una strategia comune.

cari colleghi, come ho avuto modo di affermare in sede di illustrazione della mozione, la questione della riforma della rete consolare non può prescindere da una revisione completa di tutto il panorama degli strumenti di rappresentanza degli italiani all'estero di cui dispongono il nostro ordinamento ed il nostro sistema culturale e sociale.

del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Alfredo Mantica, in merito alla prima illustrazione degli intendimenti governativi sulle politiche per gli italiani all'estero. Il sottosegretario Mantica, affrontando il tema della rappresentanza degli italiani nel mondo, ha messo in rilievo la necessità di una fattiva collaborazione tra Parlamento e Governo per una revisione delle strutture di rappresentanza esistenti per gli italiani all'estero. Il rappresentante del Governo ha anche posto ai membri del Parlamento il quesito se il ruolo dei tradizionali organi di rappresentanza, ovvero il Consiglio generale degli italiani all'estero e i Comitati degli italiani all'estero (rispettivamente CGIE e Comites), possa essere mantenuto invariato in presenza di parlamentari nazionali eletti dalle comunità all'estero. Secondo quanto affermato dal sottosegretario Mantica, a tale quesito l'orientamento del Governo è di rispondere negativamente, affrontando in Parlamento la la prospettiva di una riforma. Ecco colleghi, l'Italia dei Valori questa sfida di dare un nuovo ordine ed una nuova forma al sistema della rappresentanza, anche proponendo coraggiosi interventi, l'ha accolta ed espressa nel disegno di legge che si trova in discussione in Commissione esteri. In tale disegno di legge, che porta la mia firma, la proposta, in tre parole, è quella di sopprimere il Consiglio generale degli Italiani all'estero e di distribuire le poche funzioni che ancora il CGIE esercita in esclusiva fra i Comites, i consolati e i parlamentari eletti all'estero, ottenendo in tale modo un ampio risparmio di risorse pubbliche. Per questo ritengo che la discussione di oggi, che tratta nello specifico della riforma della rete consolare, non possa che beneficiare del contributo dato dal Parlamento e formalizzato negli impegni al Governo contenuti nelle mozioni e, dall'altra, non possa tralasciare tutto il complesso di riforma della rappresentanza, che passa dai Comites, dal CGIE e dai parlamentari eletti all'estero. Vorrei quindi darvi maggiormente conto di come, come linea dell'Italia dei Valori, i consolati rappresentino una risorsa fondamentale che non può venire sacrificata, quando invece tagli e razionalizzazioni delle risorse potrebbero avvenire su un altro organismo, ossia il CGIE. La principale ragione che mi induce a sostenere che, per molti aspetti, le funzioni assegnate al CGIE nel 1989 sono ormai state sussunte da altri organismi di rappresentanza è l'istituzione della circoscrizione Estero, con la quale si è eliminata una disparità di trattamento dei diritti dei nostri cittadini che si protraeva dalla nascita della Repubblica. In particolare, con l'elezione dei rappresentanti parlamentari dei cittadini italiani residenti all'estero, vengono ad essere assorbite tutte quelle funzioni di "consulenza" del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero, le quali, a seguito della riforma elettorale, appaiono realizzate dalla figura del parlamentare. Per ciò che concerne invece le altre funzioni che la legge n. 368 del 1989 affida al CGIE, ossia le competenze maggiormente finalizzate allo sviluppo delle potenzialità a livello locale delle comunità italiane nel mondo, ritengo, che le stesse esigenze locali

Questi, infatti, oltre ad essere più vicini alla popolazione poiché composti da membri eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero, hanno anche compiti sostanzialmente identici, come si legge nelle due leggi istitutive degli organismi. I comitati, infatti, contribuiscono, attraverso studi e ricerche, ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento, propongono e attuano iniziative in merito, riservando particolare cura alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, e intrattengono rapporti di collaborazione con i sindacati e la stampa locale. Ecco dunque che, rispetto a mantenere in piedi due enti che costano e che svolgono praticamente le stesse funzioni, abbiamo preferito, come Italia dei valori, sopprimerne uno e potenziare l'altro, perché adesso, con questo sovrapporsi di funzioni, Presidente e Sottosegretario, la situazione è un po' quella di avere doppie spese per un unico obiettivo. È come chiedere, per esempio, alla mia amica Claudia, che è avvocato, di seguire la stessa causa di Tizio e di Caio per raggiungere lo stesso risultato: se questo non è uno spreco di denaro ditelo voi. Ecco perché nella nostra proposta di legge se da una parte si abolisce il CGIE, dall'altra i comitati vengono rafforzati, facendone, ancora di più, il perno gravitazionale, a livello locale, delle multiple istanze provenienti dalle comunità degli italiani, tramite la razionalizzazione nella distribuzione dei Comites, permettendo la loro istituzione non più in base al numero di cittadini residenti, ma introducendo una criterio qualitativo che valuti davvero la realtà economica, politica e geografica locale; il potenziamento delle funzioni, dando loro una funzione di consulenza normativa in materia di iniziative legislative o amministrative e anche di accordi internazionali che interessano le comunità italiane all'estero; la previsione di meccanismi per aumentare la trasparenza e la responsabilità dei comitati nei confronti degli elettori, ponendo l'obbligo, in capo all'organismo, di redigere una relazione annuale da trasmettere al Ministro degli affari esteri, su cui discutere in Parlamento. In tale quadro, onorevoli senatori, viene da sé che il ruolo dell'autorità consolare deve accrescersi, anche grazie al rapporto di collaborazione da instaurarsi con i Comites. Il tandem fra le due strutture dovrebbe concretizzarsi sia nella predisposizione delle relazioni annuali da presentare al Ministero degli esteri che nell'individuazione delle iniziative attinenti alla vita sociale e culturale delle comunità italiane residenti nella circoscrizione consolare che, infine, per ciò che attiene la sfera economica, nell'attività di formazione professionale e di sostegno alle imprese italiane. Ma i consolati appaiono anche fondamentali nel consentire un flusso costante di informazioni tra le realtà locali estere e lo Stato italiano, le Regioni e gli enti locali. Per questo nel disegno di legge dell'Italia dei Valori si prevedono riunioni congiunte fra l'autorità consolare ed i Comites per ciò che attiene alla tutela dei diritti civili degli italiani all'estero, l'osservanza dei contratti di lavoro e l'erogazione delle provvidenze accordate, le eventuali violazioni di norme locali o europee che danneggino i cittadini italiani, le quali devono appunto essere segnalate dai Comites al consolato affinché questo si attivi presso gli organi nazionali del nostro Paese per consentire una giusta tutela o un giusto ristoro degli interessi lesi dei compatrioti residenti all'estero. proprio in considerazione della complessiva riforma che come Italia dei Valori riteniamo fondamentale per adeguare il sistema della rappresentanza all'evolversi del fenomeno migratorio italiano, mutato sia come zone geografiche di destinazione del flusso, sia come natura della migrazione, sia in termini delle esigenze che questa nuova emigrazione avverte, procedere ad una soppressione di 18 sedi consolari, alla chiusura di 2 ambasciate e al declassamento di 4 consolati generali potrebbe essere un grave errore se non viene affiancato anche da un'attività propositiva. Tale iniziativa può concretizzarsi può concretizzarsi magari tramite l'apertura di altre sedi consolari in Paesi di crescente interesse, come l'Africa, esempio tramite l'accelerazione dell'informatizzazione delle procedure, ma certamente anche attraverso una riforma del sistema Comites, parlamentari eletti all'estero e CGIE. nasce l'esigenza di illustrarvi la nostra posizione in merito al CGIE. Infatti, il futuro dei 184 Paesi in cui è presente la diplomazia italiana e di quelli in cui è invece assente (come ad esempio il Gambia, dove forse una nostra rappresentanza diplomatica potrebbe aiutare un Paese che soffre della dittatura instauratasi diversi anni fa) non può prescindere anche dalle altre forme di rappresentanza e dalle risorse che una loro semplificazione, per non dire cancellazione, Risorse che potrebbero essere impiegate non solo nella rete consolare, ma anche in istituti di cultura, scuole italiane, associazioni professionali e di categoria che operano all'estero. ribadite anche dal Governo, per la comunità italiana che vive e lavora fuori dai confini nazionali, ossia l'insegnamento della lingua italiana, l'assistenza agli italiani indigenti e il funzionamento degli organi di rappresentanza, non possono essere conseguite profìcuamente se non vengono prese in considerazione nel loro complesso.

Signor Presidente, il quadro ieri rappresentato dal senatore Micheloni mostra come sia necessario dare continuità e formalità ad un tavolo interistituzionale di confronto. Quello che sta accadendo in modo pacifico a Coira, in Svizzera, è solo uno degli indicatori della difficoltà da parte dei nostri connazionali di essere ascoltati e del timore che possano passare sulle loro teste decisioni non sufficientemente meditate e comprensibili, come pure l'indicatore di quanto sia forte l'attaccamento alle strutture consolari da parte dei nostri connazionali, ma anche delle autorità locali. Parlare di razionalizzazione e non di riforma trasmette l'idea di smantellamento, di scelta al ribasso e crea confusione anche nei ruoli, tra i cittadini, l'Esecutivo e gli eletti. La discussione avviata a seguito della presentazione del piano della rete delle sedi consolari e le reazioni determinate ci consentono però oggi di riallineare i tempi e le modalità del piano stesso iscrivendolo in un progetto più complessivo di riorganizzazione della rete che il ministro Frattini si è impegnato a presentare nel mese di gennaio. Dopo la ripetuta contrazione delle risorse sia umane che finanziarie perpetrata al sistema consolare, questo ulteriore colpo di scure ai servizi rischia veramente di compromettere non tanto l'oggi quanto la prospettiva del sistema. Vi sono infatti nei consolati situazioni molto diversificate in termini di accessibilità, ma anche di tipologia dei servizi che si sono modellate alle singole comunità. Nessuno qui oggi può negare la necessità di intervenire al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie; ne sono consapevoli anche i nostri connazionali, che però continuano ad avere bisogni sempre più diversificati, come pure diversificate sono le esigenze delle nostre imprese se vogliono utilizzare questa come rete di rappresentanza e di sviluppo della propria attività. E poiché si stanno già sperimentando forme più evolute di erogazione delle risposte, rendiamone coerente e progressiva la diffusione, come si fa in qualsiasi piano di ristrutturazione dei comparti della pubblica amministrazione, avendo ben chiaro però quale sia l'obiettivo finale, che deve essere il servizio erogato e non il mantenimento della burocrazia. È necessario quindi recuperare anche qui la logica riformista, che deve caratterizzare questo momento storico e sociale di così profondo cambiamento e che rappresenta una sfida che ci deve proiettare ad un tempo che non è domani, ma è di medio-lungo termine. Non si può quindi pensare di andare più veloci sgonfiando le ruote ad un'automobile che è già vecchia. I cittadini non sono preoccupati, Sottosegretario, di perdere burocrazia: sono preoccupati di perdere servizi o di perderne l'accessibilità. Con una popolazione anziana, qual è buona parte della nostra emigrata, l'accessibilità agli sportelli consolari diventa la condizione di utilizzo del servizio stesso. È questa l'occasione quindi di introdurre anche in tale sistema modelli più flessibili, seguendo quella logica della semplificazione che nelle parti più evolute del nostro Paese si è già radicata. Le tecnologie permettono di concentrare la produzione dei servizi, ma di mantenere anche una buona distribuzione territoriale, che è la vera garanzia per l'accesso. Più sportelli quindi e meno apparati: questa è la sfida che dovremo affrontare per costruire una rete all'altezza di un Paese che vuole giocare un ruolo internazionale di primo piano. La rete consolare rappresenta infatti l'Italia dal punto di vista sia istituzionale che amministrativo, ed è al tempo stesso l'ossatura del legame con i nostri connazionali. La strada intrapresa negli ultimi anni ha fortemente rafforzato il legame tra gli italiani nel mondo e la madrepatria. I sistemi di rappresentanza locale e parlamentare hanno di fatto formalizzato il riconoscimento di questa come la ventunesima regione, composta da quasi cinque milioni di cittadini distribuiti su cinque continenti, che sono i terminali e le antenne del nostro Paese nella globalità. E nella globalità bisogna agire avendo ben chiaro da dove si parte e dove si vuole arrivare, in una prospettiva che non può non essere che di medio e lungo termine. Il ruolo del Parlamento è quindi quello di partecipare alla definizione dei confini della delega a questa che deve essere una riforma e non un piano di emergenza e su questa il Parlamento deve esprimersi; si deve parlare di piani e non solo di tagli, di miglioramento della macchina e non di contrazione dell'offerta, di alleggerimento della burocrazia e di investimenti in formazione e tecnologia, intervenendo in quelle situazioni che oggi rischiano il congestionamento. Un esempio per tutti è l'America latina, ove giace oltre un milione di richieste di cittadinanza per le quali oggi vengono fissati gli incontri al 2013 e dove mancano persino risorse per l'invio dei plichi consolari. Anche di questo bisogna tener conto, altrimenti si fa veramente fatica a credere che dietro ci sia un obiettivo di costruzione di una rete efficiente. Lo sforzo che viene chiesto al Governo oggi in quest'Aula è quindi quello di esprimere un parere favorevole alla richiesta di sospensione di decisioni che siano definitive ed inappellabili. Ci sono oggi tutte le condizioni per procedere ad un percorso che sia condiviso, come deve essere ogni processo riformatore, che sia compreso dai cittadini nel rispetto delle proprie rappresentanze e che sia credibile per la stessa amministrazione, valorizzando anche il ruolo di tutte le componenti coinvolte. esteri*. Signor Presidente, ringrazio i presentatori delle mozioni perché offrono l'occasione di allargare il dibattito e il confronto che il Governo ha già avuto avuto sia alla Camera che al Senato nelle competenti sedi delle Commissioni esteri. Cercherò di rispondere alle varie osservazioni espresse nella discussione generale, soprattutto contribuendo alla definizione di quello che deve essere inteso come termine di confronto.

di indicare delle chiusure sapendo perfettamente che queste ultime sono la parte che più ferisce; diversamente, se avesse cominciato a parlare, ad esempio, di servizi consolari a distanza e di uso dei *personal computer*, credo che la cosa non avrebbe appassionato nessuno e non si sarebbe aperto un dibattito politico,

e nemmeno un patronato nazionale: ha un altro ruolo. Per l'assistenza, il conforto, l'aiuto, la consulenza esistono strutture che conoscete meglio di me; il consolato ha altri ruoli ed altre funzioni

mi auguro fra un po' di giudicarlo ben riuscito - per la trasformazione del Ministero degli affari esteri che, nel mondo delle tecnologie, forse cambia come sostanza (non credo che più nessuno immagini la feluca che porta ancora una lettera al Governo

su un'eventuale riforma del Ministero - il compito di rappresentare il sistema Italia nel suo complesso, rispettando il decentramento, che non è solo formale. Ad esempio, l'esistenza, l'attività ed il ruolo delle Regioni nella politica estera

in Aula per ringraziare il Comitato ristretto della Commissione esteri - di unificare intorno ad un progetto di legge in gran parte condiviso, almeno nel suo sistema di architettura portante,

alla luce delle innovazioni e delle novità in qualche modo convenute con l'elezione dei rappresentanti degli italiani all'estero.

stiamo parlando di un servizio che un cittadino italiano chiede una volta ogni dieci anni. Forse una volta ogni dieci anni si possono anche percorrere 50 chilometri di autostrada per andare al consolato più vicino!

e all'accusa di voler risparmiare sulle sedi (non so per fare quali altre cose), i Governi italiani ed il sistema Italia rispondono fornendo tale

parliamo della riforma che abbiamo visto a Bruxelles nell'ambito dei consolati; di servizi di sportello polifunzionali legati a strumenti informatici;

diritto utenti futuri di questi servizi che certamente l'Unione europea metterà in movimento. Allo stesso modo, alcuni Paesi europei - e cito la Repubblica federale tedesca - stanno avviando procedimenti di modifica dei loro sistemi sistemi di anagrafe per consentire, attraverso un documento, di riconoscere al cittadino tedesco il ruolo di cittadino europeo: dunque, un documento che viene automaticamente riconosciuto all'interno dell'Unione europea. Ma parliamo anche di cittadinanza,

cittadinanza. È stata fatta in passato, con orgoglio, perché era il recupero a questa comunità nazionale di molti cittadini italiani che avevano perso la cittadinanza nel tempo. Ma i tempi sono anche cambiati ed è trascorso abbastanza tempo per renderci conto che facciamo parte di un sistema europeo, nel quale la nostra regola di legge e di cittadinanza è assolutamente anomala e anormale. Credo che tutti voi sappiate che in Spagna esistono molti cittadini italiani di origini argentina che sono cittadini italiani per la legge italiana e che, nella stessa loro condizione, un cittadino spagnolo residente in Argentina non sarebbe mai un cittadino spagnolo.

e gli esponenti politici italiani; o nel luogo di residenza come cittadini italiani residenti all'estero, ma anche come cittadini europei per le liste e i candidati che in quel Paese si presentano al Parlamento europeo; o nel modello che definisco di "sezione elettorale condominiale", cioè portando sempre un'urna,

Ecco, l'insieme del confronto e del dialogo, che diventa politico perché molti di questi temi ovviamente sono politici, sebbene nei fatti e nel concreto si misurino in sedi, uffici, impiegati, ruoli,

A Saarbrücken esistono due consolati generali: uno è quello nostro, per il quale parliamo di chiusura, e l'altro è quello francese. Peraltro, ricordo agli immemori che la Francia confina con la Saar. Il consolato di Francia è titolato consolato generale, ma tutti sappiamo che in realtà è un ufficio di rappresentanza. Allora, fare di Saarbrücken

Siccome non credo che il senatore Micheloni volesse intendere questo, vorrei che, per lo meno sul piano dell'onestà intellettuale, non si partisse ponendo paletti di questo tipo, perché allora l'avventura sarebbe estremamente difficile e pericolosa.

Su tutto questo, con grande sensibilità e grande disponibilità da parte di tutti, ci stiamo avviando a definire in qualche modo qualcosa di nuovo, di innovativo, non solo in termini di reti diplomatiche e consolari ma anche di rapporti tra Governo e Parlamento, rispettando quella che era - credo - la missione strategica indicata dall'onorevole Mirko Tremaglia, che qui voglio ringraziare e di cui sono l'indegno erede, anche perché mi tocca in qualche modo cercare di avviare o modificare molte delle cose che lui aveva costruito nel tempo ma che erano a quel tempo assolutamente necessarie e fondamentali.

«impegna il Governo: ad approfondire il progetto di riordino della rete degli uffici all'estero, non tralasciando l'altrettanto necessaria rivisitazione dei compiti e delle funzioni delle numerose istituzioni che oggi rappresentano ed operano in favore dei cittadini italiani all'estero; a ripensare al progetto di riordino delle istituzioni sopra citate tenendo presente: *a)* l'importanza strategica di taluni uffici di rappresentanza del nostro Paese all'estero; *b)* l'imprescindibile ruolo delle nuove tecnologie nel processo di ammodernamento delle procedure amministrative; *c)* il necessario e costruttivo confronto con il Parlamento».

la sede competente delle Commissioni affari esteri per contribuire all'analisi delle iniziative di razionalizzazione degli uffici diplomatici e consolari; ad avviare quanto prima un confronto con le Commissioni parlamentari competenti per una valutazione strategica del ruolo della rete degli uffici all'estero».

propostaci dal sottosegretario Mantica. Con la discussione svoltasi oggi, credo che ci si sia proposti non soltanto di avviare riforme istituzionali ovvero organizzative, ma ma che si sia parimenti toccato le urgenze ed i bisogni essenziali degli italiani all'estero, ricordando allo Stato il dovere, prima di tutto morale, di assicurare una vita dignitosa anche ai suoi cittadini residenti in altri Paesi. Garantire l'assistenza sanitaria, tramite interventi strutturali sulle necessità locali come in Colombia, Venezuela o Argentina; permettere 1'estensione dell'assegno sociale erogato dall'INPS alle categorie disagiate anche ai cittadini italiani indigenti residenti all'estero; o ancora consentire ai loro figli di imparare la lingua italiana, o infine dare a tutti coloro che vivono all'estero il diritto di votare, tutti questi aspetti importantissimi dipendono anche dalla creazione di una struttura consolare efficiente e capace di intervenire concretamente nella vita di chi, italiano per cultura storia e origine, si trova momentaneamente o stabilmente all'estero. La rete diplomatica infatti è fondamentale non solo nelle relazioni internazionali, ossia per mantenere i rapporti bilaterali con gli altri Paesi o sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo, ma ha anche ma ha anche il ruolo imprescindibile di perseguire finalità solidaristiche per gli italiani che vivono all'estero. Perché non dobbiamo dimenticarci, cari colleghi, che se il fenomeno degli emigrati italiani

del nostro Stato. Auspico che fra le questioni da prendere in analisi ci sia anche quella concernente un altro tipo di migrazione. Mi riferisco alla migrazione dei giovani che si muovono sul territorio comunitario ed extracomunitario non per fame come i loro nonni, ma per fama, ossia per la ricerca di esperienze che ne qualifichino i *curricula* e per tirocini di formazione.

il possibile scontro interculturale con la pratica di vita quotidiana, non vengano attratti da altri sistemi nazionali dove è più semplice trovar lavoro o costruire famiglia, ma possano diventare «profeti in patria propria». L'impegno a cui si richiama il Governo con la mozione dell'Italia dei Valori non è quindi soltanto quello di formulare politiche e normative che sappiano razionalizzare le risorse che spendiamo per la rappresentanza consolare, ma anche quello di creare una rete diplomatica che possa incrementare le condizioni di vita degli italiani espatriati nei loro Paesi di accoglienza, i quali risultano essere più di 4 milioni, rendendo l'Italia il Paese con il più alto numero di cittadini residenti all'estero. E il dovere statale di tutelarli non è sostenuto solo dal nostro partito, ma trova una fonte altissima anche nella Convenzione internazionale sui lavoratori migranti, adottata dalle Nazioni Unite nel 1990. Per ciò che riguarda la riforma della rete consolare - lo abbiamo già detto - poiché la la rete diplomatico-consolare rappresenta il punto di contatto tra i cittadini italiani all'estero e lo Stato italiano, per quanto attiene sia alla rappresentanza che ai servizi e alla tutela internazionale; e poiché tale rete è stata più volta sottoposta a riduzione dei capitoli di bilancio relativi al suo funzionamento, sia nelle ultime finanziare che nelle manovre aggiuntive e di assestamento di bilancio, siamo convinti che ogni ipotesi di riorganizzazione della rete consolare non deve tradursi in chiusura di consolati, o riduzione di personale, o meno diritti per il personale. Allo stesso tempo riteniamo che le soluzioni debbono comunque essere individuate con il metodo della concertazione, come chiede anche come chiede anche il SNDMAE, il sindacato a cui è iscritta la stragrande maggioranza dei diplomatici italiani. Ecco perché nella mozione chiediamo di ripensare di ripensare al progetto di riordino tenendo presente l'importanza strategica di taluni uffici di rappresentanza del nostro Paese all'estero, l'imprescindibile ruolo delle nuove tecnologie e il necessario e costruttivo confronto con il Parlamento. Cari colleghi, è proprio in questa sede, è proprio in questa sede, infatti, che devono essere individuati i contenuti dei progetti di riorganizzazione e razionalizzazione, che vanno da una riforma del sistema Comites-CGIE, sopprimendo gli enti doppione, ad una maggiore assistenza agli istituti di cultura e alle scuole di italiano, fino ad una valorizzazione del ruolo del parlamentare eletto all'estero. Auspico davvero che il Governo sappia tenere in considerazione le mozioni di cui si discute oggi, nonché la risoluzione dell'onorevole Narducci approvata alla Camera il 21 luglio scorso che anche noi dell'Italia dei Valori abbiamo condiviso, e tutte quelle reazioni di forte perplessità fra i cittadini e le autorità locali che la manovra di razionalizzazione della rete consolare annunciata dal Governo ha suscitato. Di un indebolimento del sistema consolare, infatti, ne potrebbero risentire non solo i cittadini italiani residenti all'estero, con le loro esigenze e i loro legittimi diritti, ma anche economicamente le imprese italiane, il turismo verso l'Italia, nonché in generale lo *status* del nostro Paese nel mondo. Oltretutto, i risparmi derivanti dalla manovra di razionalizzazione così come comunicati dal Governo - sarebbero davvero di poco conto. Infatti, non sono stati quantificati i costi veramente notevoli derivanti dal trasferimento di strutture e personale, e non è stato dato conto da parte del Governo di quanto invece si potrebbe conseguire con una concreta lotta agli sprechi o con una semplificazione delle procedure, che forse permetterebbe di spendere meno, fare di più e di non dover chiudere ‑ lo ripeto ancora una volta - ben 18 consolati e 2 ambasciate. In conclusione, voglio soltanto dire che se - come me - pensate che gli italiani che risiedono fuori dai confini nazionali non rappresentino una semplice appendice del popolo italiano ma siano una risorsa fondamentale; se ritenete - come me - che siano gli ambasciatori

anche dolorosa ma sicuramente doverosa, che non si consegue tramite un taglio alle ambasciate ma attraverso un progetto di riforma che abbraccia tutti gli organismi di rappresentanza, Comites e CGIE *in primis.* una riforma che si interroga su quali siano le esigenze della nuova forma di emigrazione e cerca di rispondervi concretamente in ottica "*glocal*", quella cioè per la quale occorre agire localmente per conseguire risultati globali. globali. Concludo affermando che bisogna disegnare un quadro efficiente, volto al risparmio, agevole e capace di stabilire un dialogo permanente tra comitati di base, consolati, parlamentari e Ministro degli esteri, perché si allarghino davvero i confini dell'Italia: e non parlo di quelli geografici, ma di confini umani. Cari colleghi, è questo il motivo per cui vi chiedo di votare favorevolmente la mozione dell'Italia dei Valori, che è cosciente della assoluta necessità di razionalizzare le risorse pubbliche, in quanto mai come oggi l'esigenza di ridurre le spese pubbliche è sentita dai cittadini e richiesta dalle istituzioni comunitarie; mai come oggi una ristrutturazione che snellisca l'apparato burocratico è vissuta come fondamentale dagli attori coinvolti. Presidente, onorevoli senatori, signor sottosegretario Mantica, è già a partire dall'inizio degli anni Novanta che la rete diplomatico- consolare del nostro Paese è stata sottoposta ad un procedimento progressivo di ristrutturazione. Tale procedimento, forse non sempre equilibrato e coerente, si è tuttavia evidenziato come sempre più necessario sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, tanto da essere rilanciato con molta forza

illustrateci chiaramente nel giugno scorso e oggi dal sottosegretario Mantica, che ci ha proposto un piano ampio e rigoroso, pur mostrando disponibilità a discutere ed ascoltare le sollecitazioni che immagino, cari colleghi, anche voi, come me, ricevete quotidianamente da parte dei nostri connazionali residenti in ogni parte del mondo. Partiamo dalla consapevolezza, condivisa in questa Assemblea, che le modalità organizzative ed il *modus operandi* delle rappresentanze italiane possano e debbano essere migliorate, razionalizzando le spese e offrendo un servizio più efficiente e più mirato sia per i concittadini residenti fuori dal Paese sia per gli operatori italiani che guardano oltre frontiera. Ben venga dunque la digitalizzazione dei servizi, soprattutto nelle aree dove l'informatizzazione e i servizi di connettività sono diffusi e largamente accessibili. Tutta l'area europea e nordamericana devono essere dotate al più presto, secondo noi, degli strumenti per svolgere in via telematica, e per quanto possibile anche a domicilio, le funzioni amministrative ed il rilascio di attestati e documenti, compatibilmente, come è ovvio, con il livello più alto di sicurezza del trattamento dei dati personali. La chiusura ed il ridimensionamento delle sedi, che merita sicuramente una mappatura accurata e ragionata e che deve passare attraverso la consultazione dei cittadini italiani residenti nelle varie aree, è tuttavia un sacrificio necessario. Dobbiamo renderci conto che la rete consolare non è da concepirsi come "struttura" ma come "servizio", come elemento, cioè, dinamico e non statico, reattivo rispetto alle evoluzioni delle dinamiche della politica estera e commerciale e pronto ad adeguarsi all'innovazione tecnologica ed ai vantaggi, di tempo, di costo, di capillarità, che essa può offrire. La diplomazia segue oggi canali molteplici ed impensabili rispetto a pochi decenni fa.

la Lega Nord propone da tempo un rafforzamento di altre funzioni, in particolare quelle di supporto agli operatori economici. Oggi il pluralismo dei soggetti (rappresentanze diplomatiche, istituto per il commercio estero, camere di commercio, istituti di cultura), che faticano a parlare con una voce sola, rischia di indebolire l'immagine del Paese, di generare contraddizioni, di lasciare anelli deboli e dunque, in sostanza, di non sfruttare appieno le potenzialità della presenza italiana nel mondo. Credo che puntando su una sinergia vera tra questi enti sia possibile, a parità o anche con minori risorse, se necessario, ottenere risultati buoni e soprattutto costituire un punto di riferimento forte per tutti gli operatori italiani ed un interlocutore autorevole per i partner locali. Spero dunque che anche il dibattito su questa mozione si inserisca nella discussione che abbiamo iniziato in Parlamento in chiave costruttiva perché la riorganizzazione avvenga sulla base di decisioni condivise affinché esse si rivelino opportune e durature,

*(PD)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, sottosegretario Mantica, senatrici e senatori, mi limiterò ad una panoramica necessariamente rapida sui punti salienti della mozione di cui è primo firmatario il senatore Micheloni, riservandomi di consegnare il testo integrale dell'intervento qualora non rientrassi nei limiti di tempo concessimi. Mi consenta, signor Presidente, in primo luogo di esprimere il mio rammarico per la vistosa assenza, quasi totale, dei colleghi della maggioranza. *(Applausi

Se noi pensiamo all'Aula parlamentare come ad un Consiglio comunale, è ovvio allora che l'obiezione è giusta. Ma è molto più ricco, più denso e più completo il processo democratico. Quindi, non accediamo a queste critiche da antipolitica;

senatori, gli elementi portanti di questa mozione sono essenzialmente due: valutare la portata, la correttezza di modalità e sufficienza di analisi, l'impatto sui settori di politica estera e politica economica, oltre che sulle politiche per gli italiani nel mondo, della decisione del Ministero degli affari esteri di sopprimere 18 sedi consolari (13 in Europa, 2 negli Stati Uniti, 2 in Australia, 1 in Africa) e declassare 4 Consolati generali; avviare un confronto in sede parlamentare sulla razionalizzazione della rete diplomatica e consolare, in modo da verificarne i criteri di necessità ed equità, La chiusura di una sede consolare non comporta solo la scomparsa di un ufficio di servizi, informazione, rappresentanza. Prelude, già nel medio e breve termine sul territorio dove l'ufficio è insediato, ad effetti negativi a cascata. Scompare un punto di riferimento, un erogatore di servizi, un motore di iniziative, un testimone visibile e palpabile d'italianità per le comunità, sia di cittadini italiani che di cittadini del Paese ospitante. La trasmissione di lingua e cultura perde di stimolo, controllo, richiamo. Le Camere di commercio italiane, dove ci sono, e ce ne sono in molte aree del mondo come attesta l'attività di coordinamento, indirizzo, raccordo e promozione dell'Assocamere estero, dell'Assocamere estero, non hanno più *in loco* un sostegno istituzionale. L'immagine dell'Italia si distorce e sfoca. Con la chiusura di un consolato muore un pezzo d'Italia nel mondo. E il tutto - questa cosiddetta "razionalizzazione" della rete consolare che va anche sotto il nome di "accorpamenti" - con il vago obiettivo di risparmiare la miseria di 8 milioni di euro (bruscolini nel contesto del bilancio pubblico) quando la riforma-sfascio dovrebbe andare a pieno regime nel 2011. Un risparmio molto dubbio. Appena pochi Appena pochi giorni fa, il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, Giacomo Sanfelice di Monteforte, ha testualmente dichiarato in merito: «Il risparmio non è la nostra stella polare». Per forza non ci sarà risparmio. Per forza. Mentre si scandiscono i nomi delle città del mondo con le due prime dozzine di tradizionali consolati da sopprimere, sono ancora in fase di prima sperimentazione, se non addirittura di progettazione, varie formule di spersonalizzazione nel servizio pubblico, gli sportelli consolari permanenti al posto degli uffici soppressi, le postazioni di rilevamento delle impronte digitali da aprire all'estero per il passaporto biometrico. Una benissimo tutto quanto le innovazioni tecnologiche nelle comunicazioni possono offrire per migliorare i servizi dell'Italia nel mondo. Ma vorrà venire qualcuno a spiegarci, dati alla mano, perché nella fase di passaggio alle "magnifiche sorti e progressive", una fase che sarà di anni e forse anche di decenni, si debbano azzerare postazioni dell'Italia all'estero, dove il calore e le capacità del rapporto umano diretto costituiscono ancora, e continueranno a costituire per tempi indefinibili, la base di un autentico servizio personale al gruppo etnico italiano espatriato o oriundo, uno strumento ausiliare dell'internazionalizzazione degli scambi e del sistema produttivo del Paese, un aspetto rilevante di politica estera e di politica culturale? Altri colleghi che rappresentano nelle nostre Aule parlamentari la circoscrizione elettorale Estero saranno più competenti e aggiornati di me ad illustrare la situazione nelle loro specifiche ripartizioni dell'Europa e dell'America settentrionale toccate dalla soppressione di sedi consolari. Più direttamente, in veste di eletto nella ripartizione Oceania-Africa-Asia, mi preme sottolineare la situazione che viene a determinarsi con l'annunciata chiusura dei consolati di Adelaide e Brisbane in Australia e di Durban in Sud Africa. Si intende privare di una rappresentanza ufficiale italiana un'area di oltre 4 milioni di chilometri quadrati, il 60 per cento dell'intero continente australiano. Dovrebbe andare soppresso il consolato di Brisbane, capitale dello Stato del Queensland, con giurisdizione anche sul Northern territory, con capitale Darwin: in tutto oltre 3 milioni di chilometri quadrati, con una forte presenza storica di cittadini e oriundi italiani. Dovrebbe sparire anche il consolato ad Adelaide, capitale dello Stato del South Australia: 985 mila chilometri quadrati, equivalente a tre volte l'Italia. Ora riflettiamo sulla "razionalità" degli accorpamenti prospettati in Australia. Le pratiche del consolato di Brisbane dovrebbero passare a Sydney, 730 chilometri a sud e un'ora e mezzo di volo; quelle di Darwin a Perth, 4.040 chilometri ad ovest e oltre quattro ore di volo; quelle di Adelaide a Melbourne, 654 chilometri a est e un'ora di volo. Mi permetto di ricordare, rispetto a quanto detto dal senatore Mantica, che si tratta di distanze ben

una città dove non solo risiedono 4.000 cittadini italiani e altrettanti, se non più, oriundi, ma che è anche lo scalo marittimo e lo snodo commerciale più importante dell'intero continente africano; la città dove si registra la massiccia presenza di aziende italiane con un giro di affari, in appalti, prodotti e servizi, di oltre 300 milioni di euro; dove attraccano 50 navi italiane all'anno, in pratica una a settimana, con relativa richiesta di assistenza consolare per il disbrigo di pratiche di navigazione; dove la sola *Mediterranean Shipping Company* impiega in pianta stabile 300 cittadini italiani. Per tornare all'Australia, ad Adelaide e Brisbane sono state raccolte 15.000 firme - non poche centinaia - per una petizione al Ministro degli affari esteri italiano, con l'appello a soprassedere alla chiusura di quei due consolati. Un'intera seduta del Parlamento del South Australia è stata dedicata alla «decisione romana» - così viene chiamata - con appelli a ripensamenti e l'accusa di colpo basso alla grande comunità italiana di quello Stato e all'intero ospitale popolo sudaustraliano. Hanno scritto direttamente al presidente del consiglio Berlusconi i *premier* dello Stato del South Australia, Mike Rann, e del Queensland, Anna Bligh. I quotidiani australiani hanno pubblicato una dichiarazione del primo ministro federale Kevin Rudd, il quale, in un incontro privato a margine del G8 dell'Aquila, avrebbe ottenuto l'impegno di Berlusconi ad intervenire sul disegno di chiusura dei consolati in Australia. Anche il "Forum dei parlamentari italo-australiani", al quale aderiscono 40 componenti di nascita o origine italiana delle legislature federale e regionali d'Australia, ha fatto pervenire sulla questione un messaggio al presidente Berlusconi. Quando si arriva al punto in cui Governi e Parlamenti di Paesi esteri, legati da tradizionali vincoli d'amicizia all'Italia, si sentono in dovere di intervenire sulla chiusura di rappresentanze consolari sui loro territori, allora non si è più di fronte ad una semplice e ordinaria decisione amministrativa interna del Ministero degli affari esteri, bensì ad una situazione dai ben più ampi e delicati risvolti di relazioni internazionali che impattano sull'immagine e gli interessi del nostro Paese all'estero e che meritano un franco ed esauriente confronto in sede parlamentare. Per queste ragioni, il Gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto favorevole alla mozione.

ci indica che la maniera di condurre la politica estera nell'epoca in cui viviamo è fondamentalmente cambiata, o sta cambiando velocemente, rispetto al *modus* tradizionale di condurre la politica estera e di valorizzare ciò che questa tradizionalmente metteva in rilievo. Credo che i rapporti mutati tra gli Stati, il ruolo delle organizzazioni internazionali, il procedere della storia implichino anche un nuovo o rinnovato modo di condurre la politica estera. oggi si trattano accordi attraverso contatti bilaterali fra i Capi di Stato; lo fanno la Francia e la Germania, lo sta facendo il nostro Paese e lo fanno naturalmente gli Stati Uniti, cioè quegli Stati che hanno un regime presidenziale o che hanno affidato un primo modo di condurre la politica che noi non conoscevamo nel passato. Così come la stessa figura dell'ambasciatore, oggi rivestita anche di un ruolo manageriale oltre che diplomatico-rappresentativo,

di rappresentanza all'estero conta 122 ambasciate, 110 consolati, 89 istituti di cultura, 117 uffici dell'ICE, 140 camere di commercio, 24 uffici ENIT e qualche altra rappresentanza che probabilmente mi sfugge o sfugge alle classifiche. Questo sistema necessita di una razionalizzazione che risponde appunto a quelle nuove esigenze di cui parlavo e non soltanto, come il Sottosegretario ha appena detto, a logiche di restrizione finanziaria o a problemi amministrativi e burocratici. Il Sottosegretario ha illustrato il modo con cui il Governo intende procedere a questa razionalizzazione; ha parlato di interventi modulati nel tempo,

la fitta trama delle associazioni fra sindacati e patronati, i parlamentari eletti all'estero; tutte figure, istituzioni, organizzazioni che portano avanti le stesse istanze di rappresentanza sociale dei nostri cittadini. Non mi sembra

a sostituire tale quadro di rappresentanza sociale con un sistema elettoralistico costruito attorno alla figura del candidato al Parlamento, come è stato detto nell'ultima assemblea del CGIE: mi sembra

al concetto di democrazia contemporanea. Contrariamente a quanto avviene in Italia, dove ormai la possibilità di partecipare alla dinamica democratica è totalmente cancellata dalla vigente legge elettorale, i collegi esteri offrono ancora

Abbiamo dedicato un paio di ore per cercare di affrontare una questione che, come giustamente ricordava il sottosegretario Mantica, non dovrà cambiare a seconda del colore della parte politica che governa. Tuttavia la

ed alcuni rappresentanti del Gruppo Misto, votare qualcosa sul quale il Governo ha espresso il suo parere favorevole. È vero che il Presidente del Consiglio vorrebbe che i rappresentanti dei Gruppi votassero per tutto il Gruppo, magari aggravando le caratteristiche della non democrazia contemporanea, però questa sarà sicuramente l'ultima volta in cui non parteciperò a un voto. Dalla prossima volta, come abbiamo iniziato a fare con i trattati internazionali, toccherà chiedere il voto elettronico per cercare di limitare la deriva della democrazia contemporanea, tanto cara al nostro Presidente.

può obbligare all'ascolto chi non può intervenire partecipando? Come vede, è un tema di grande sostanza. Se chi ascolta può intervenire, è ovvio che partecipa, perché partecipa del processo decisionale, ma se lei vuole obbligare un collega

Chi non può intervenire, ovviamente non può essere obbligato ad ascoltare, e questo mi pare ovvio. Se uno invece può intervenire, allora è chiaro il suo riferimento, senatore Perduca, ed ha ragione, perché se posso intervenire nel dibattito, posso alzare la mano e parlare. e parlare. Se non vengo, vuol dire che non dimostro interesse e non svolgo quella che è una mia opportunità e un mio compito. Tuttavia, obbligare chi non può intervenire ad ascoltare in Aula e non nel suo ufficio, oppure, ad esempio, a non ascoltarla con tanto interesse su Radio radicale non mi sembra una cosa interessante.*(Commenti

Prima di procedere alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Io avevo proposto di aggiungere anche i Comitati competenti delle Camere, anche questi in sede congiunta. Posso capire la reazione del sottosegretario Mantica, e quindi non formalizzo tale richiesta; vorrei ricordare a me stesso e ai colleghi l'esistenza del Comitato per le questioni degli italiani all'estero e non di una Giunta che avrebbe risposto

Presidente, mi conceda di ringraziare tutti i senatori che hanno partecipato al dibattito, di ringraziare anche i pochi colleghi presenti in modo concreto, non virtuale, e di ringraziare gli innumerevoli virtuali che sicuramente hanno seguito con attenzione il nostro dibattito.

al concetto della non partecipazione alle sedute.

effetti questa mozione ci dà modo di trattare un tema di non secondaria importanza nel richiamare il Governo agli impegni che ha assunto nell'ambito della Convenzione internazionale sull'aiuto alimentare. l'ONU ha stabilito nell'assemblea del 2000 che entro il 2015 dovremmo raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione della fame nei Paesi poveri, nei Paesi in via di sviluppo. È chiaro, quindi, che la fame è una delle grandi questioni globali, che toccano l'uomo, che toccano l'ambiente, che toccano il nostro stesso futuro, futuro che non è più relegato ormai alla comunità locale o all'attenzione al nostro piccolo, ma ad un futuro che attraversando noi stessi e le nostre famiglie ci collega al mondo.

di incontri tra Paesi industrializzati a cerchio più o meno allargato e di dibattiti molto importanti. Spesso queste grandi conferenze si esauriscono in dibattiti non concludenti, che evidenziano sempre di più la spaccatura esistente tra un mondo oramai considerato sviluppato, anche se alla ricerca di una sua identità nell'era postmoderna,

della legislazione dei singoli Stati. Forse, per scarso impegno o disinteresse, forse perché tutti noi anche in quest'Aula siamo condizionati dall'emergenza dell'oggi che ci sovrasta e magari non ci si accorge che questa stessa urgenza è determinata proprio dalla distrazione rispetto alle suddette grandi questioni globali, questioni globali, che non richiedono la fretta dell'oggi quanto piuttosto uno sguardo più lungo per essere affrontate e magari ci aiuterebbero poi a risolvere implicitamente anche tanti problemi dell'oggi. la grande questione ambientale. Al riguardo è in corso la Conferenza di Copenaghen per riscrivere il Protocollo di Kyoto. Vi è poi il problema di riscrivere le regole dei mercati di finanza, vale a dire il tema della redistribuzione della ricchezza nel mondo.

Si calcola che vi sia circa un miliardo di vittime della fame, a cui se ne aggiungono ogni anno circa 100 milioni. Un numero impressionante che, tra l'altro, non si sta riducendo, ma sta crescendo. In altri termini, c'è un'enorme parte del mondo in cui la globalizzazione sta aggiungendo danni a danni e che è esclusa da qualsiasi forma di sviluppo. Paesi in cui la fame e la malattia sono endemiche e fanno ancora milioni di vittime. Paesi in cui vi è la preoccupazione della sopravvivenza più elementare che impedisce la promozione dell'uomo nella sua integralità. E quando parlo di promozione

se non l'indicazione di un obiettivo, come recita anche l'ultima enciclica del Papa, «*Caritas in veritate*»", cioè far uscire i popoli dalla fame, dalla miseria, delle malattie endemiche e dall'analfabetismo? Questo è il vero obiettivo dello sviluppo. le condizioni in cui il male, nelle sue diverse articolazioni, può facilmente attecchire e albergare: guerre fratricide e tribali, fanatismi religiosi, la stessa schiavitù. È straordinario come in alcuni Paesi non si riesca a portare riso, grano, alimenti ma, in compenso, si riescano ad introdurre armi; qui l'obiettivo della modernità è semplicemente la sostituzione delle frecce con le pallottole. veramente non credo sia degno di un Paese o di una civiltà moderni. Ed è ipocrita non accorgersi di questi fenomeni, così come è ipocrita non rendersi conto che gran parte dei fenomeni migratori di cui discutiamo quotidianamente in Aula sono dovuti a tali condizioni di miseria. Se, quindi, non aiutiamo questi popoli ad uscire da condizioni di sottosviluppo, non riusciremo a creare le condizioni per una minima stabilità globale che ci permettano davvero di lavorare su un progetto di progresso civile e, quindi, di uscire dalla paura. Se non lavoriamo su questo grande progetto globale, la post-modernità rischia di perpetuare le sue incertezze. Se non riusciamo ad agganciare allo sviluppo globale quella metà del mondo che oggi ne è esclusa, la globalità non sarà rosea. Ci si prospettano due scenari: possiamo aver un mondo più unito, più stabile, più ricco, con mercati più aperti, più pulito e più solidale, ovvero possiamo consegnare al futuro un mondo più cupo, più egoista, chiuso, conflittuale, fatto di comunità il lotta tra loro per una sopravvivenza migliore.

e per conseguirlo appare prioritario il diritto all'alimentazione. La fame, come riconosciuto anche dal recente Vertice FAO, non è solo frutto di una scarsità materiale, ma soprattutto frutto di una scarsità sociale, su cui dobbiamo lavorare. Ed è una scarsità di natura innanzitutto istituzionale. Le crisi alimentari sono spesso provocate da atti di irresponsabilità politica, nazionale o internazionale, frutto di Governi che si preoccupano del proprio arricchimento, e che fanno della corruzione e della violenza strumenti di governo quotidiano del Paese. Vi è un interesse da parte di alcuni Governi al mantenimento delle popolazioni in condizioni di indigenza o di guerra perpetua, per garantire al regime autoritario la propria sopravvivenza. Su questo tema politico insieme agli aiuti alimentari dobbiamo ragionare fortemente perché, ripeto, la fame è spesso il frutto di un'emergenza sociale e politica.

questioni legate al mercato comune. Non si riesce a creare una condizione di multilateralità, di promozione di tecniche agricole ed industriali, di dimensionamento delle riserve e delle risorse locali. Per citare ancora l'enciclica, la via solidaristica allo sviluppo dei Paesi poveri può costituire un progetto di soluzione nella crisi globale in atto; e sottolineo la parola solidarietà, che declina in termini politici la fraternità. fraternità. Non è scontata, oggi, la solidarietà, partecipa poco al nostro dibattito politico, ed io la contrappongo in qualche modo alla cultura secolare alla cultura secolare a cui forse attribuiamo l'incertezza, l'insicurezza che stiamo vivendo, questa debolezza d'identità dell'Europa che fa aumentare gli egoismi, le paure, che ci fa ripiegare su noi stessi invece di promuovere le migliori capacità; questa debolezza intrinseca che non ci fa capire che oggi siamo cittadini del mondo. Tutto ciò è attribuito alla cultura secolare che stiamo vivendo: ma cos'è la cultura secolare se non, probabilmente, la mancanza di una cultura politica vera, di riferimenti politici veri, l'insufficienza che culture politiche come il socialismo e in parte anche il liberalismo hanno prodotto nella società globale non riuscendo più a dare risposte? Allora, se parliamo di società solidale, il primo punto è rispettare gli impegni. In un'ottica solidale, gli impegni non devono essere traditi, altrimenti il risultato è peggiore

aiuto solidale per alleviare il problema della fame nel mondo, con un impegno di 200 milioni di euro accumulato dal 2003 ad oggi, che vede l'Italia in ritardo rispetto ai *partner* internazionali. È un problema di dignità e di coerenza del mio e nostro Paese di fronte ad un milione di persone che muoiono di fame. è un problema quindi di credibilità: non potremo affrontare grandi problemi se prima non riusciamo ad assumere, nel piccolo, le nostre responsabilità per affrontare la prima emergenza umanitaria che è la morte per fame nel mondo.

con la mozione che il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato intendiamo chiedere al Governo, ancora una volta, di dare finalmente seguito, in maniera concreta, agli impegni che più volte sono stati assunti dal nostro Paese in sede internazionale, in relazione al contrasto alla fame nel mondo, adottando un'azione forte di difesa del diritto al cibo, al fine di arginare l'emergenza alimentare dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo. Il Governo italiano si deve impegnare a far sì che la lotta alla povertà e lo sviluppo agricolo rimangano al centro dell'agenda politica sia nazionale sia internazionale e che la sicurezza alimentare, con particolare riferimento all'Africa, rimanga una delle priorità dell'agenda politica mondiale, concretizzando un impegno forte a livello globale e azioni reali da parte di tutta la comunità internazionale. L'ultimo rapporto della FAO sull'insicurezza alimentare nel mondo denuncia che oggi sono quasi un miliardo le persone che soffrono la fame, quasi un sesto della popolazione mondiale. Secondo la FAO la sicurezza alimentare dovrà necessariamente diventare la priorità dell'agenda politica mondiale. Il Vertice FAO, svoltosi recentemente a Roma, ha confermato gli impegni della vigilia. Almeno a parole: i 192 Paesi dell'ONU dichiarano di voler rafforzare gli sforzi per dimezzare il numero degli affamati entro il 2015. I mezzi finanziari per raggiungere in così poco tempo questo obiettivo, già di per sé irrealistico viste le cifre spaventose di coloro che soffrono la fame, non sono indicati. L'impegno c'è, i finanziamenti purtroppo no. Per nutrire circa un miliardo di persone affamate non bastano i buoni propositi: il mondo ha bisogno di decisioni politiche concrete e di risorse ben investite. Eppure, come ha spiegato anche il Papa intervenendo al Vertice FAO, oggi il mondo produce il cibo necessario per sfamare tutti: la terra è in grado di nutrire sufficientemente tutti i suoi abitanti. Infatti, se equamente distribuita, la produzione attuale è in grado di garantire cibo anche ai 900 milioni di esseri umani cronicamente malnutriti che tuttavia, in modo sistematico, non riescono ad essere sfamati. Allo stato attuale dunque, il problema non è da ricercarsi nella scarsità della produzione alimentare quanto piuttosto nel limite all'accesso agli alimenti da parte delle persone più povere. L'abisso che separa i più ricchi fra i ricchi dai più poveri fra i poveri è diventato infinitamente più profondo: un mondo paradisiaco per alcuni e infernale per i più, dove le cento persone più ricche del pianeta hanno una fortuna superiore a tutto ciò che possiedono un miliardo e mezzo di abitanti messi insieme. La povertà suscita ancora commiserazione ma sempre meno indignazione; si continua a diffondere l'idea che i poveri sono il risultato del caso o il frutto della fatalità, ma mai quello di precise scelte politiche dì governi che, con l'indifferenza o talvolta la complicità della comunità internazionale, annientano la dignità, assieme alla vita, di milioni di esseri umani. Dunque, il problema della fame è soprattutto un problema di povertà e di ingiustizia sociale. E non è un caso se le maggiori preoccupazioni attengono proprio al futuro. Da un lato, la popolazione mondiale sta continuando a crescere anche se con una velocità minore rispetto al passato e, dall'altro, c'è una forte quanto preoccupante caduta di investimenti nella ricerca agricola che rischia di condizionare la capacità di sviluppo della produzione alimentare futura. L'attuale crisi finanziaria in atto ha avuto qualche ripercussione anche sul minore impegno dei Paesi ricchi nel contrasto alla fame nel mondo, ma purtroppo il calo di attenzione da parte dei Paesi ricchi nei confronti della lotta alla fame nel mondo non è una questione di oggi. Un esempio al riguardo è offerto dai negoziati commerciali multilaterali della *World trade organization* (WTO) che vanno sotto il nome di Doha Round; il negoziato, partito nel 2001, è ormai bloccato da anni, perché non c'è alcuna disponibilità da parte dei Paesi industrializzati a fare concessioni rispetto alle richieste dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo. Anche se occorre distinguere le posizioni in campo. L'atteggiamento dell'Unione europea è stato finora più responsabile anche perché la riforma della Politica agricola comune è andata nella direzione di ridurre le distorsioni in essere a cominciare, ad esempio, dall'eliminazione dei sussidi all'esportazione e dalla riduzione dei sussidi interni. Finora, come Unione europea, abbiamo realizzato molte iniziative: ne è un esempio la Convenzione sull'aiuto alimentare, firmata a Londra il 13 aprile 1999, che si propone come finalità il conseguimento della sicurezza alimentare nel mondo e il miglioramento della capacità della comunità internazionale di poter far fronte a situazioni di emergenza alimentare e di sopperire al fabbisogno alimentare dei Paesi in via di sviluppo. L'Italia ha aderito e dato esecuzione alla suddetta Convenzione con la legge 29 dicembre 2000, n. 413, attraverso la quale sono stati stanziati 36,2 milioni 36,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 ed è stato affidato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) l'incarico di provvedere all'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo mediante la fornitura a questi ultimi della quota di partecipazione italiana. Il Comitato per l'aiuto alimentare - organo istituito dalla Convenzione sull'aiuto alimentare dell'Accordo internazionale sui cereali del 1967 composto da tutte le parti della Convenzione di Londra e responsabile della sua applicazione - ha più volte prorogato, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione, la Convenzione medesima. La legge 17 giugno 2004, n. 155, ha quindi autorizzato la spesa di 36,2 milioni di euro per l'anno 2003, accumulando un primo ritardo di oltre un anno rispetto agli impegni assunti, mentre l'articolo 5*-bis* del decreto-legge n. 182 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, ha stabilito che fossero stanziati solo 18,1 milioni di euro (invece dei 36,2 previsti per l'anno di competenza), dunque per il solo primo trimestre del 2004. Il nostro Paese, a seguito della decisione - adottata nel novembre 2005 dal III Governo Berlusconi - di dimezzare i fondi precedentemente stanziati per far fronte agli adempimenti derivanti dalla adesione a detta Convenzione sull'aiuto alimentare, risulta inadempiente per quasi 200 milioni di euro e rischia perciò l'esclusione dalla stessa. Siamo quindi fermamente convinti che l'adesione dell'Italia alla Convenzione ed i relativi impegni finanziari per ottemperare a quanto in essa stabilito darebbero modo al nostro Paese di giocare un ruolo strategico al fianco delle maggiori potenze industrializzate del mondo, nella politica di sicurezza alimentare in favore dei Paesi in via di sviluppo. Pertanto, è necessario che il nostro Paese provveda a sanare immediatamente la situazione di inadempienza nei confronti della Convenzione di Londra sugli aiuti alimentari, ottemperando - così come chiesto anche dai colleghi del PD con PD con la loro mozione - all'impegno finanziario connesso alla partecipazione dello Stato italiano alla Convenzione sull'aiuto alimentare e impegnandosi concretamente nella lotta contro la fame nel mondo. Con la nostra mozione vogliamo altresì richiamare l'attenzione del Governo sull'importanza che assume - così come ormai riconosciuto da tutti gli Stati e da tutti gli organismi internazionali e sovranazionali un corretto rapporto con le organizzazioni non governative, al fine di realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ed in considerazione del loro ruolo essenziale nell'attuazione degli interventi di emergenza e, più in generale, nel settore delle iniziative riguardanti la sicurezza alimentare e la lotta alla malnutrizione. Accanto alla difesa del diritto al cibo e al perseguimento dell'obiettivo di sconfiggere la fame nel mondo entro il 2015 come previsto dalla stessa Dichiarazione del Millennio, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 2000 - vogliamo chiedere altresì al Governo un impegno a promuovere un'azione diplomatica efficace, tramite la nostra rappresentanza diplomatica all'ONU, in relazione ad una riforma della FAO che rappresenta una delle principali organizzazioni internazionali del settore, al fine di consentire un migliore e più efficace funzionamento nell'interesse dei Paesi più poveri del mondo.

È questo un problema regolamentare, su come funziona il Parlamento, oppure no? Attendo risposta e passo ora all'intervento. In questo clima, appunto, intimo vorrei far presente che la mozione in esame, che era nata prima del G8 e prima del Vertice FAO, ci ricorda che un miliardo di persone soffrono la fame nel mondo. Non è un caso. Un miliardo e 400 milioni di persone vivono con meno di un dollaro al giorno. Non è un caso. Il reddito nazionale lordo dei 49 Paesi più poveri è inferiore al reddito delle tre persone più ricche del mondo. Non è un caso.

che questi impegni non sono stati mantenuti; che la cooperazione allo sviluppo, in un discorso più generale, ha subìto tagli più alti dei denari che sono rimasti; che la legge sulla cooperazione allo sviluppo non è stata fatta nonostante si fosse arrivati ad un testo unico; che era stato promesso dal ministro degli affari esteri Frattini che, dopo il G8, sarebbe sta nominato un responsabile della cooperazione nel nostro Paese.

È evidente che il dibattito sulla fame nel mondo avrebbe avuto bisogno di una presenza, diciamo, meno virtuale, anche considerando il nostro pessimo risultato

Lo sappiamo anche noi che abbiamo presentato questa mozione che le risorse non bastano mai e che le necessità sono grandi e quant'altro. Vorrei però dire al collega Quagliariello - che ogni volta che parla ci dà lezioni di catechismo che andrebbero fatte in altri luoghi

è pensabile governare un mondo in cui il 20 per cento delle persone consuma l'80 per cento delle risorse? È pensabile governare con una variante degradante del capitalismo che si chiama capitalismo consumista? Diciamolo ancora, in queste Aule, che noi viviamo secondo un sistema che non funziona, che non va bene; che - forse siamo rimasti in pochi a pensarlo - non esiste il pensiero unico; che la fine della storia non è avvenuta, come diceva Fukuyama; che forse è il caso di ripensare il sistema,

come sia possibile che nel 2008 i raccolti di cereali siano cresciuti del 4,9 per cento, raggiungendo l'ammontare *record* di 2.230 milioni di tonnellate (pari ad un chilo al giorno per ogni essere umano)

Poiché è quel che è dato in comune per l'uso di tutti ciò che tu ti annetti. La terra è data a tutti e non solamente ai ricchi». Signora Presidente, il dibattito che oggi svolgiamo avviene all'immediato indomani del Vertice della FAO a Roma e durante il Vertice sul clima a Copenhagen:

dibattito, muoiono per fame più di 300 bambini. Alla fine di questa giornata ne saranno morti più di 17.000: 6.000.000 di persone ogni anno ancora muoiono per fame nel nostro pianeta. Sono passati nove anni dai solenni impegni assunti dal Vertice del Millennio, come ci ha ricordato il senatore Bosone: l'obiettivo così ambizioso di dimezzare il numero delle persone che soffrono la fame. Un obiettivo che resta lontanissimo; anzi, il numero delle persone che nel mondo sono condannate alla fame ha ricominciato a crescere. Posso usare qui le parole con cui il nostro Presidente del Consiglio ha aperto il mese scorso il Vertice mondiale mondiale sulla sicurezza alimentare a Roma. Succede così raramente che posso essere d'accordo con il Presidente del Consiglio che voglio utilizzare l'occasione. Ha detto il Presidente del Consiglio: «Negli ultimi due anni le conseguenze della crisi (finanziaria, economica e sociale) sui poveri del pianeta sono state pesantissime. Ogni mese si sono aggiunti sette milioni di poveri agli 850 milioni tra uomini, donne e bambini che già si trovano in una condizione di denutrizione. Si è raggiunto così il massimo storico di oltre un miliardo di persone affamate (...)». Perché? Perché la recessione economica globale si è aggiunta alla crisi alimentare ed energetica, limitando i redditi e le opportunità di lavoro per i poveri del mondo e perciò le opportunità di accesso al cibo. Questa è naturalmente una mia considerazione. Dobbiamo avere consapevolezza delle cause, lo hanno ricordato i colleghi. Il problema non è quello di una scarsa offerta alimentare mondiale (il senatore Di Giovan Paolo ci ha ricordato che anche il 2009 vi è stata una produzione agricola sui livelli *record* del 2008): il problema è la forte speculazione sui prezzi delle derrate alimentari. Comunque, a fine 2008 i prodotti alimentari domestici costavano il 25 per cento in più di due anni prima e questo significa per centinaia di migliaia di persone passare da uno stato di sopravvivenza all'assoluta impossibilità di sopravvivere. Una fonte non sospetta, «L'Osservatore Romano», ci segnala che il 70 per cento delle transazioni, causa dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari, sono di natura finanziaria, cioè speculazione sulle *commodity* alimentari. è poi il problema di una globalità della crisi che ha colpito contemporaneamente vaste aree del globo. Vi è il problema di una riduzione degli investimenti esteri (si calcola circa un terzo). Vi è una riduzione soprattutto delle rimesse degli emigrati. Attenzione: noi discutiamo tanto dal punto di vista nostro interno, ma come è stato per la storia del nostro Paese (prima abbiamo parlato dei nostri consolati all'estero a sostegno della vita dei cittadini italiani),

Diminuisce - si stima - di circa un quarto l'assistenza allo sviluppo per i 71 Paesi più poveri. Allora, noi prendiamo molti, moltissimi impegni diciamo, belle parole nei Vertici internazionali: resta il fatto che, a due terzi del percorso dell'impegno così rilevante di diminuire della metà la fame nel mondo, essa aumenta e purtroppo non è diminuita.

dei Paesi donatori: ebbene, l'Italia si colloca purtroppo al 21° posto su 23 Stati e abbiamo perso due posizioni negli ultimi due anni. Dietro di noi restano solo il Portogallo e la Grecia. E tra gli elementi che ci fanno collocare così indietro nella graduatoria vi è proprio la divaricazione tra gli impegni che assumiamo e l'incapacità di mantenerli. Io naturalmente voterò a favore anche di questo aumento del contingente italiano in Afghanistan, però è intollerabile che quando si tratta di mandare soldati rispondiamo in tre giorni e quando si tratta di onorare gli impegni di una cooperazione internazionale più capace di cambiare le cose non bastano gli anni per adempiere agli impegni. *(Applausi dal Gruppo* *PD)*. Ricordiamo qui la situazione della Convenzione sulla sicurezza alimentare. Siamo inadempienti dal 2003 e per questa parte c'è una responsabilità condivisa dei Governi che si sono succeduti. Con quale credibilità, chiedo al Governo e a noi stessi,

aumentati. Abbiamo sottoscritto impegni per fondi aggiuntivi per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria, ma come facciamo a sostenere questi fondi se non ce ne sono di nuovi e più che dimezziamo quelli che erano disponibili? 321 milioni di euro significa il 56 per cento in meno di quelli - già pochi - esistenti nell'anno precedente, il minimo dal 2000. Ormai la cooperazione raccoglie più soldi dalle fonti private (400 milioni di euro) di quanto dia lo Stato (321 milioni di euro).

sottosegretario Mantica, anche una figuraccia in Europa, perché l'Europa non riuscirà a raggiungere il*target* dello 0,56 per cento proprio perché l'Italia non onora i suoi impegni. Credo che manchi, come osservano le associazioni che rappresentano le ONG italiane che agiscono nel campo della cooperazione internazionale, la disponibilità nel fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze per finanziare i fondi delle banche regionali di sviluppo, rendendo perciò impossibile l'erogazione dei contributi che fanno capo a impegni pregressi; tanto meno riusciremo a onorare i nuovi impegni che abbiamo assunto. Questi sono, purtroppo, dei fatti.

siano cose che non servono più. Occorre il coraggio dei fatti e sapere che anche gli interessi nazionali si difendono meglio se abbiamo il coraggio di cambiare questo stato di cose.

esteri*. Signora Presidente, devo dire che rispondere in pochi minuti agli appassionati interventi di oggi è estremamente difficile,

Però su qualche punto credo vada fatta almeno una valutazione di carattere generale. In Italia - è stato detto anche recentemente da tempo la cooperazione incide sempre meno sul prodotto interno lordo; cioè diminuisce sostanzialmente la capacità di fare cooperazione da parte del nostro Paese. Questa è una riflessione talmente vera che è radicata in un arco di tempo di ormai 16 anni.

questo radicamento. Lo 0,2 per cento del PIL in realtà non è mai stato superato in questi 16 anni, e la tendenza è addirittura a diminuire; di questo, in occasione della scorsa legislatura, quando si è parlato di riforma della cooperazione, si è molto discusso. Credo discusso. Credo vi sia da parte di tutti gli operatori, di tutte le forze politiche e sociali e delle organizzazioni non governative, la necessità di fare un salto di qualità quando si affronta tale argomento. Cioè, ragioniamo troppo spesso in termini di una liberalità dei Paesi ricchi nei confronti dei Paesi poveri, come se una quota parte del nostro reddito, quella che grosso modo fa parte della voce "regali", sia quella da destinare agli impegni di cooperazione. Non entriamo nell'ordine di idee che l'aiuto allo sviluppo è un investimento e, come dire, un modo per essere nelle relazioni internazionali, per creare condizioni diverse e difendere il nostro stesso interesse nazionale nel quadro di un equilibrato sviluppo del mondo; restiamo al concetto di liberalità e lo gonfiamo ancor di più nella logica solidaristica estrema, per cui alla fine questo dono - l'ho detto più volte quando ero responsabile della cooperazione - gratifica il donatore ma molto spesso non interessa colui che lo riceve, un dono che viene fatto nella logica del donatore. Ecco, questo credo sia un tema culturalmente profondo su cui occorre un impegno e un dibattito serio, perché temo che, se non si esce da questa logica in un momento in cui la crisi finanziaria è aumentata, e aumenta quindi la pressione sui conti ordinari dello Stato, di dibattiti come quello di questa mattina potremmo farne

Ora, anche questo è un altro equivoco che esiste nella struttura istituzionale del nostro Paese, perché non è vero che la cooperazione del Ministero degli affari esteri sia la cabina di regia o l'elemento determinante della politica di cooperazione e aiuto allo sviluppo.

di intervento sull'Unione europea, perché, evidentemente, non è nemmeno corretto parlare oggi di cooperazione italiana allo sviluppo dimenticando che una cifra ormai molto significativa (più del doppio di quello che il Governo italiano nella sua autonomia può spendere) viene spesa attraverso l'Unione europea.

volta, i potenti della Terra - uso questa espressione che nel dibattito di oggi mi piace - si incontrarono con cinque grandi Capi di Stato africani, a cominciare dal presidente della Repubblica sudafricana Mbeki,

alle ragioni per cui ciò è avvenuto, certo non c'è stata da parte di nessun Governo, né di centrodestra né di centrosinistra, una determinata volontà per cambiare la situazione, ma tecnicamente vorrei ricordare che non a caso gli intervenuti hanno ricordato, anno per anno,

affari esteri. Verifico in quest'Aula, insieme ai colleghi parlamentari, che la tabella A del Ministero degli affari esteri è una delle cose con cui più ci si diverte quando

il reperimento dei fondi per rispondere alla Convenzione di Londra, per la quale per ogni anno occorre comunque approvare un provvedimento legislativo, mancano 270 milioni di euro.

segue: «a colmare con la necessaria gradualità dettata da esigenze di rigore finanziario l'arretrato dell'Italia nei confronti della sopra citata Convenzione di Londra sugli aiuti alimentari; a perseguire concretamente l'obiettivo della sicurezza alimentare nel mondo, sostenendo tutte le iniziative promosse dalle Nazioni unite per l'agricoltura e l'alimentazione;

volta al raggiungimento dell'obiettivo di sconfiggere la fame nel mondo, come previsto dalla Dichiarazione (...), se occorre prendendo in considerazione proposte di riforma degli organismi internazionali preposti alla lotta contro la fame nel mondo».

in un'azione, attraverso la sua rappresentanza diplomatica all'ONU, per una nuova prospettiva di funzionamento dell'inefficace FAO perché ciò evidentemente non è, nelle relazioni esterne, diplomaticamente accettabile.

per le questioni degli italiani all'estero, ho partecipato al Vertice della FAO sulla sicurezza alimentare mondiale. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, ha dato il via ai lavori con una frase capace di colpire le coscienze di tutti noi. Oggi la faccio mia inizio la mia dichiarazione di voto citandolo: «Alla fine di questa giornata» - ha affermato Ban Ki-Moon - «quando saremo ancora qui, oltre 17.000 bambini saranno morti di fame. Ne scompare uno ogni cinque secondi. Ne scompare uno ogni cinque secondi. Sei milioni in un anno». Colleghi, circa 24.000 persone muoiono ogni giorno per fame o cause ad essa correlate e tre quarti di questi decessi interessano bambini di età inferiore ai cinque Oggi, nel 2009, il 10 per cento dei bambini che vivono in Paesi in via di sviluppo muoiono prima di aver compiuto i cinque anni. Il problema della malnutrizione non si misura, solo attraverso il numero dei decessi. Oltre alla morte, la malnutrizione cronica provoca uno stato permanente di affaticamento che causa una bassa capacità di concentrarsi e lavorare, un'estrema suscettibilità alle malattie e un generale indebolimento della vista. Viene stimato che a soffrire di malnutrizione siano 800 milioni di persone, ovvero 100 volte il numero di persone che effettivamente ne muoiono ogni anno. Cari colleghi, di fronte a queste cifre non si può, né tanto meno si deve rimanere inerti. Come saprete, il nostro Paese con la legge 29 dicembre 2000, n. 413, ha ratificato la Convenzione sull'aiuto alimentare, siglata a Londra il 13 aprile dello stesso anno. Tale Convenzione, che si compone di un preambolo e di 27 articoli, ha lo scopo di contribuire a fronteggiare i problemi di sicurezza alimentare a livello mondiale, con particolare attenzione ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo. Nel testo vengono specificate le quantità annuali minime per le quali i membri si impegnano e sotto quale forma tali aiuti possano essere essere forniti. Nello specifico, i Paesi contraenti possono scegliere se donare prodotti alimentari o denaro finalizzato all'acquisto di questi ultimi, se vendere provvigioni contro moneta del Paese beneficiario o se, infine, vendere prodotti alimentari a credito, rimborsabile in modo scaglionato su periodi di 20 anni o più e a tassi inferiori a quelli commerciali internazionali. La Convenzione, così come ratificata nel 1999, prevedeva, infine, all'articolo 25, che la stessa, in vigore fino al 30 giugno 2009, potesse essere prorogata oltre tale data dal Comitato di aiuto alimentare per periodi consecutivi di non più di due anni.

18,1 milioni di euro, in grado dunque di coprire solo il saldo relativo al primo semestre del 2004. Oltre all'esclusione dalla Convenzione, l'Italia rischia di trovarsi in difficoltà all'interno dell'Unione europea.

presentata, ha affermato che, a causa delle esigue risorse disponibili presso il Fondo speciale del Ministero degli esteri, il Ministro degli esteri non ha potuto presentare un provvedimento sulla materia. Vista l'entità della cifra dovuta non è possibile immaginare nemmeno, a detta del Sottosegretario, un ricorso ai fondi ordinari della cooperazione. Altro fatto grave è che la stessa Craxi, ammettendo l'insufficienza della risposta, abbia cercato di rassicurare l'elettorato e i deputati presenti in Aula, ricordando l'iniziativa per la sicurezza alimentare globale lanciata dal Governo in ambito G8. In realtà, cari colleghi, leggendo il documento conclusivo del *Summit* dell'Aquila, si legge che i grandi della terra hanno sì deciso di mobilitare nei prossimi tre anni 20 miliardi di dollari in favore degli agricoltori dei Paesi poveri, soprattutto africani, al fine di promuovere lo sviluppo rurale e l'autosufficienza, ma lo hanno fatto senza specificare in che modo gli Stati partecipanti al Vertice intendano reperire e garantire questi fondi. qui non si tratta di dover aderire o meno a questa Convenzione. L'allora Governo e le Camere hanno già discusso in merito. Oggi si tratta di dar fede all'impegno assunto ed è vergognoso evitare di affrontare il tema e ancora più grave assumere nuovi impegni. sesto anno di vita. Questi non sono solo dei fallimenti a livello internazionale. Sono dei fallimenti anche per noi, noi singoli Stati e singole Nazioni. che si sta diffondendo a livello internazionale non è positivo. È un virus che va combattuto e lo si può debellare solo se crediamo negli impegni che i nostri Esecutivi assumono. In conclusione, cari colleghi, vorrei ricordarvi l'importanza della collaborazione internazionale in materia di cooperazione allo sviluppo. Per debellare il problema della fame nel mondo non è sufficiente, infatti, che i singoli Stati stanzino aiuti e mandino, ad esempio, provvigioni di grano. Occorre bensì promuovere una crescita economica sostenibile ed equilibrata e garantire una stabilità politica nelle zone dilaniate da conflitti. Proprio per la massiccia portata di questi interventi si rende necessario collaborare e affidare questi compiti a delle organizzazioni internazionali o sovranazionali, nonché garantire loro solidi finanziamenti e il mantenimento degli impegni presi. Cari colleghi questa è la posizione dell'Italia dei Valori e mi auguro che possa essere condivisa nella maniera più trasversale possibile. Grazie.

Ci risulta estremamente difficile, infatti, non essere d'accordo sulla necessità di rafforzare l'impegno, che deve essere comune a tutti, per combattere tale fenomeno. Argomento questo che deve trovare condivisione da parte di tutti i Paesi sviluppati. Va sicuramente ricordata e evidenziata la Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare quale strumento di efficace contrasto alla fame nel mondo. È giusto ricordare che detta Convenzione è stata conclusa dalla Comunità europea con decisione n. 421 del 2000 e prorogata poi di anno in anno dal Comitato per l'aiuto alimentare per ben quattro volte, restando, di conseguenza, in vigore fino al 30 giugno 2009. Ad oggi, un'ulteriore proroga per un periodo di un anno è stata giudicata nell'interesse della Comunità, tanto è vero che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione n. 27 aprile scorso, ha autorizzato la Commissione a sostenere la necessità di detta proroga in sede di Comitato per l'aiuto alimentare. Facile quindi intuire che la questione relativa all'applicazione della Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare oggetto delle mozioni in discussione

Oltre a ciò ritengo però necessario richiamare l'attenzione riguardo alla sostanziale inadeguatezza che, negli anni, le politiche fondate sull'aiuto alimentare hanno mostrato rispetto all'obiettivo di fornire risposte serie ed efficaci al problema della fame nel mondo e della sicurezza alimentare. Nel passato, purtroppo, ci si è concentrati maggiormente in grandi dichiarazioni di intenti piuttosto che in iniziative che volevano risolvere a fondo il problema. Di conseguenza, sono convinto che non appare particolarmente corretto enfatizzare il ruolo di tali politiche, a meno che - come sembra non si vogliano utilizzare i ritardi e le disfunzioni nella loro attuazione per mettere in difficoltà il Governo. Riteniamo che affrontare il tragico problema della fame nel mondo richieda un approccio di respiro più ampio, concetto che ha trovato contrario ampia conferma nei risultati del vertice G8 svoltosi quest'anno all'Aquila, così che - come traspare dal documento ufficiale conclusivo - si è deciso di mobilitare per i prossimi tre anni una cifra ben notevole (stiamo parlando di 20 miliardi dollari) a favore degli agricoltori dei Paesi poveri, Paesi poveri, soprattutto quelli africani, per promuovere lo sviluppo rurale e l'autosufficienza alimentare. Questo impegno dimostra in maniera inequivocabile come il problema della fame nel mondo sia stato concretamente affrontato da questo Governo,

o una disponibilità di beni alimentari sufficienti, ma perché vi è un numero crescente di persone che non dispone dei mezzi economici per comprarsi da mangiare. Vorrei citare il premio Nobel Amartya Sen che, già nel 1998, ci ammoniva ricordando che «la fame è il risultato del non avere abbastanza da mangiare. Non è il risultato del non esserci abbastanza da mangiare». Ciò non è che non c'è da mangiare, ma che non possono comprarsi da mangiare, e credo che questo sia un argomento sul quale tutti quanti dobbiamo riflettere. Sul piano del problema della fame nel mondo assistiamo, invece, ad un progressivo - e questo ci deve far preoccupare - impoverimento delle popolazioni già povere e all'inevitabile aumento del numero dei sofferenti la fame, che sono passati da 844 milioni ad oltre un miliardo negli ultimi dieci anni, ossia proprio nel periodo in cui, stando ai famosi e tanto declamati del Millennio della FAO, avrebbero dovuto avviarsi verso il loro dimezzamento, che la stessa FAO aveva eannunciato per il 2015. si ritiene sufficiente evidenziare quanto le più avanzate espressioni degli attuali sistemi produttivi agro-industriali, ossia le coltivazioni transgeniche e le colture *no-food*, si siano rivelate rispettivamente poco efficaci e poco efficaci e potenzialmente pericolose rispetto alla drammatica esigenza di contrastare il problema della fame nel mondo. Le coltivazioni delle piante geneticamente modificate, dopo quasi 15 anni di produzione su larga scala, hanno evidenziato alcuni limiti rappresentati sia dal limitatissimo numero di specie coltivate - di fatto sono poche, solo soia, mais, colza e cotone - sia dall'ancor più ridotto impiego dei relativi prodotti, in larga parte destinati o alla produzione di mangimi o all'impiego in filiere agro-industriali, i cui prodotti in ogni caso non sono non sono destinati assolutamente a rispondere all'esigenza di fornire cibo alle popolazioni più povere. Le coltivazioni *no-food*, in specie quelle destinate a produrre biocarburanti, pongono il grave problema della concorrenza nell'uso di risorse, quali la terra e l'acqua, altrimenti destinabili alla produzione di cibo. Al riguardo credo corretto e sicuramente significativo ricordare che per ricordare che per produrre 100 litri di bioetanolo (ossia più o meno un pieno di carburante di un'automobile di grossa cilindrata) occorrono 236 chili di mais, quantità che, in termini di chilocalorie, corrisponde a quanto necessario per assicurare il mantenimento alimentare di un uomo per un anno. È evidente che continuare a legare le politiche per combattere la fame nel mondo alle sole misure di aiuto alimentare, sicuramente indispensabili per far fronte a situazioni di emergenza, ma del tutto insufficienti per affrontare problemi strutturali come la fame, significa chiudere gli occhi sia sia sui disastri provocati dallo scellerato liberalismo senza regole degli ultimi anni, sia sul colpevole fallimento - come hanno evidenziato anche i colleghi che mi hanno preceduto - di organismi come la FAO, che già nel 1996 si era data l'obiettivo di dimezzare il numero di persone sofferenti la fame entro il 2015. Al contrario, i risultati sono andati in modo sicuramente sicuramente diverso.

puntare sui piccoli agricoltori di quelle terre, sui giovani e sulle loro famiglie, potenziando il loro accesso alla terra, fornendo loro gli strumenti per sviluppare

Anche il Santo Padre, in occasione dell'ultimo Vertice FAO, ha dichiarato che il problema dell'insicurezza alimentare va affrontato eliminando le cause strutturali che lo provocano e promuovendo lo sviluppo agricolo dei Paesi poveri mediante investimenti in infrastrutture rurali, in sistemi di irrigazione, in trasporti, in organizzazione di mercati, in informazione e in diffusione di tecniche agricole appropriate, capaci cioè di utilizzare al meglio le risorse umane, naturali e socio-economiche maggiormente accessibili a livello locale. Occorre rafforzare il legame dell'agricoltura con i territori, con il cibo e con le tradizioni alimentari delle popolazioni interessate, affinché lo sviluppo sia il risultato della valorizzazione delle risorse endogene, umane ed ambientali, presenti a livello locale. Concludo, signor Presidente, dicendo che con questo spirito riteniamo di invitare il Governo ad impegnarsi sul fronte della lotta alla fame del mondo,

*(PD)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarazione di voto a nome del Gruppo del Partito Democratico. Naturalmente cercherò di rispettare i tempi assegnati, e per questa ragione chiedo di poter consegnare il testo integrale

è del 17 giugno scorso: questa è la ragione per cui è stata poi adeguata, diciamo attualizzata. Fu redatta in quella data e sottoscritta da molti colleghi in quanto era imminente lo svolgimento del Vertice G8 all'Aquila nel quale sarebbe stato riservato particolare spazio all'approfondimento sui temi della malnutrizione e dell'accesso al cibo. Il Partito Democratico, per la verità, già in prossimità del Vertice FAO del giugno 2008 ricordò, attraverso propri documenti e comunicati, le risultanze della Conferenza di Roma, fortemente voluta e promossa dal governo Prodi, durante la quale fu fu assunto tra l'altro un impegno concreto nei confronti del fondo fiduciario della sicurezza alimentare della FAO con uno stanziamento di 100 milioni di dollari, di cui 75,7 furono tempestivamente versati. Si trattò di un'iniziativa rilevante, che rispose positivamente all'esortazione avanzata dalla FAO ai Paesi donatori di accentuare i propri interventi di assistenza e di valutare l'opportunità di riprogrammare gli aiuti ai Paesi poveri penalizzati dal rialzo dei prezzi delle derrate. I G8 all'Aquila hanno lanciato un programma da 20 miliardi di dollari per i prossimi tre anni, salvo a definire impegni e modalità concreti non solo sul piano dell'effettivo versamento delle risorse finanziarie, ma anche, come ricordava il collega dell'indirizzo e della finalizzazione delle medesime. II recente Vertice FAO del novembre 2009 ha richiamato l'attenzione internazionale sulla necessità di dare risposte alla globalizzazione dei mercati, affidando all'agricoltura la possibilità di diventare il perno intorno al quale far crescere una politica economica mondiale, in grado di riequilibrare le sorti produttive e finanziarie dei Paesi in via di sviluppo. Il documento finale, tuttavia, non fa alcun richiamo alla richiesta del direttore generale della FAO, Jacques Diouf, di destinare 44 miliardi di dollari allo sviluppo agricolo e alle infrastrutture nei Paesi poveri, lamentando, inoltre, anche una riduzione del 22 per cento dei fondi nazionali indirizzati alla FAO e del 32 per cento di quelli relativi al personale impiegato rispetto ai livelli raggiunti nel 1994. Secondo quanto affermato dal Direttore generale della FAO bastano «44 miliardi di dollari l'anno di aiuti ufficiali allo sviluppo da investire in infrastrutture, tecnologia e moderni *input* produttivi. Questa cifra» - sono le parole dello stesso Diouf - «è ben poca cosa se paragonata ai 365 miliardi di sussidi all'agricoltura che sono stati dati ai produttori dei Paesi OCSE nel 2007 ed ai 1.340 miliardi che si sono spesi in armamenti lo stesso anno». In sostanza, si tratta di mettere a regime un sistema economico che consenta al pianeta di nutrire se stesso, o meglio i suoi abitanti più deboli, anche perché cominciano a vedersi i risultati degli sforzi compiuti da molti Paesi dell'Africa, dell'America latina e dell'Asia per ridurre il numero di persone sottonutrite. Richiamo solo per accenno il programma del Governo brasiliano lanciato nel 2003 il gruppo PD ritiene, peraltro in piena adesione alle indicazioni che emergono dal documento FAO approvato durante l'ultimo Vertice, che sia arrivato il momento di rilanciare l'agricoltura per sostenere con politiche economiche internazionali il reddito dei piccoli coltivatori ed assisterli nella qualificazione della produzione, in modo da dare anche risposte adeguate al rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari che penalizzano i consumatori poveri. È necessario, dunque, avviare una strategia che insista su più fronti al fine di produrre più cibo laddove è più urgente: adottare politiche e programmi per assicurare il sostentamento di milioni di poveri a rischio di inedia; promuovere misure per aiutare gli agricoltori dei Paesi in via di sviluppo attraverso un potenziamento della produttività e un ampliamento della produzione al fine di creare reddito e opportunità di lavoro per le popolazioni rurali povere. Il Partito Democratico ritiene che sia urgente sollecitare l'impegno della comunità internazionale in modo che il tema della sicurezza alimentare divenga parte integrante delle politiche di sostegno che i Paesi sviluppati assumono a favore dei paesi più poveri e svantaggiati. Non mi soffermerò sui dati che sono doviziosamente riportati nel corpo della mozione Bosone, che lo stesso primo firmatario ha illustrato nel suo intervento, ma è giusto che vada qui sottolineata - nell'intento di offrire attraverso l'approvazione di questa mozione un contributo serio e propositivo ad un problema così drammatico - la necessità che il Governo mantenga gli impegni assunti dallo Stato italiano per effetto della firma della Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare del 1999 e reperisca le risorse necessarie per regolare i versamenti cui si è obbligato. L'ottemperanza di tale adempimento e gli ulteriori oneri che il Paese ha assunto a seguito del G8 di L'Aquila nonché dell'ultimo vertice FAO, rappresenterebbero una risposta seppur parziale al problema, tuttavia finalmente degna di una civiltà avanzata e responsabile e di una avvertita sensibilità dinanzi al grande tema della fame nel mondo e delle disuguaglianze, sul quale il Papa Benedetto XVI ha espresso un severo monito proprio nel

Signor Presidente, abbiamo trovato, di buona intesa con la maggioranza, un punto di sintesi nella parte dispositiva del testo della mozione, naturalmente

dunque auspico che - in considerazione della straordinaria rilevanza dell'argomento in discussione - l'Aula voglia pronunciarsi unanimemente. Naturalmente preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. **Testo

le due mozioni oggetto di votazione presentate dai colleghi Bosone ed altri e Di Nardo ed altri, pur presentando reciprocamente elementi di diversità nelle premesse, nella parte dispositiva sostengono con chiara e apprezzabile univocità l'opportunità che l'Italia abbia a sostenere anche in futuro un intervento concreto nell'azione multilaterale nell'azione multilaterale per combattere la piaga dell'insufficienza alimentare mondiale, la piaga della povertà e della morte a causa della povertà. del tutto evidente che il Gruppo del PdL sostiene con la massima convinzione tale indicazione, giacché corrisponde esattamente a quanto sin qui dichiarato e fatto dal presidente del Consiglio Berlusconi e dall'intero Governo in numerose e recenti occasioni. Mi riferisco all'Aquila, ancora prima a Genova, come ha opportunamente ricordato il sottosegretario Mantica, a Cison di Valmarino, dove si è tenuto il primo G8 agricolo della storia storia e, in modo particolare, all'azione concreta, reiterata, forte, decisa, convinta e appassionata del presidente del consiglio Berlusconi, del ministro degli affari esteri Frattini, del ministro dell'agricoltura Zaia, e oggi, in Aula, del sottosegretario Mantica. Sono convinto che quanto disposto dalla Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare nel 1999 possa ritenersi sostanzialmente superato e, quindi, assorbito - così si direbbe in gergo parlamentare - dal dispositivo del G8 dell'Aquila; tanto nella sostanza, nella sostanza, l'entità degli aiuti, quanto nella forma, cioè nelle modalità di aiuto, come diceva molto opportunamente il mio collega e amico Vallardi della Lega. Come ricordato dal presidente del Consiglio Berlusconi in occasione del Vertice FAO sulla sicurezza alimentare tenutosi recentemente a Roma, «negli ultimi due anni le conseguenze della crisi finanziaria, economica e sociale sui poveri del pianeta sono state pesantissime ogni mese si sono aggiunti sette milioni di poveri agli 850 milioni tra uomini, donne e bambini che già si trovavano in una condizione di denutrizione. Si è raggiunto così il massimo storico di oltre un miliardo di persone affamate, circa 100 milioni in più rispetto al 2008». Lo stesso Capo del Governo ha sottolineato che il lavoro del *Summit* G8 dell'Aquila «ha dato frutti concreti con la dichiarazione adottata il 10 luglio scorso da oltre 40 Paesi e organismi internazionali», in cui si è messo «nero su bianco l'impegno per un fondo di 20 miliardi di dollari in tre anni».

a perseguire con strumenti adeguati l'obiettivo di garantire a centinaia di milioni di esseri umani, oltre al nutrimento, la dignità, la libertà, la speranza e - vorrei dire - anche la capacità di diventare essi stessi produttori, più solo assistiti, non solo più o meno grati, come diceva il Sottosegretario per un aiuto elargito, ma autori essi stessi della propria sopravvivenza e del proprio sviluppo. Ciò che colpisce maggiormente nel documento dell'Aquila è anche il richiamo da tutti avvertito a dover innovare per quanto riguarda le modalità di aiuto. Si tratta, infatti, di imboccare con decisione la strada che deve portare i Paesi più sviluppati a sostenere la capacità produttiva agricola locale come elemento centrale per il contrasto alla sottoalimentazione, per combattere la povertà, per fornire elementi di speranza a popolazioni disperate, per tentare di arginare o comunque moderare i fenomeni di massiva emigrazione, diversamente assolutamente incontrollabili. Quindi, non è solo nostro dovere, è anche nostro interesse farlo ed anche in fretta e bene. Volendo solo per un attimo entrare nel dettaglio delle questioni rilevate nelle due mozioni, ricordo che la situazione emergenziale legata al problema della fame nel mondo ha portato alla Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare del 1999, già ben delineata, che ha istituzionalizzato l'aiuto alimentare in favore delle popolazioni più povere inserendolo in un contesto normativo comune a tutti i Paesi aderenti, che si sono impegnati a fornire ai Paesi in via di sviluppo un aiuto alimentare

che porterebbe ad un valore del grano oggi di 317 euro la tonnellata. Ora, sappiamo tutti che se i contadini italiani potessero percepire dalla vendita del proprio grano 317 euro alla tonnellata farebbero voti a tutti i Santi, a quelli che sono stati ricordati prima dal collega Di Giovan Paolo ma anche a tutti gli altri che non sono stati ricordati. Sappiamo tutti che la

quindi circa un terzo rispetto a quanto disposto nei parametri, ripeto sballati, di Londra.

non ho bisogno di ricordarmelo troppo per la verità) che negli ultimi due anni abbiamo assistito in Italia, in Europa e nel mondo ad una caduta verticale delle quotazioni dei cereali ad una caduta verticale delle quotazioni delle *commodities* agricole, della soia, del mais, del frumento tenero, del frumento duro, dell'ordine del 40-50 Ricordo a me stesso che nel 1979 il prezzo della soia in Italia era di 79.000 lire al quintale; oggi siamo a 32 euro il quintale. siamo di fronte a fenomeni di questo tipo: nel medio periodo, negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad una caduta verticale dei prezzi. C'è stata un'impennata per fenomeni speculativi due anni fa, ma è un po' come un elettrocardiogramma impazzito,

si trovano una situazione di povertà; ovviamente, non una povertà paragonabile a quell'altra povertà di cui stiamo discorrendo, però in una situazione di grave difficoltà. Vado a concludere,

che ha portato entrambi i Gruppi proponenti a volerle modificare, attualizzare, ed anche disporre in maniera tale che il Governo potesse accoglierle.

Ormai abbiamo di fronte a noi degli obiettivi ben più ambiziosi che dobbiamo assolutamente mantenere fermi: non solo perché ne siamo convinti, non solo perché è giusto, non solo perché è un problema di uguaglianza e di sviluppo, ma perché ci conviene. Noi, ricchi del mondo occidentale ricco, con tutte le sue povertà e con tutte le sue miserie, abbiamo tutto l'interesse ad arrivare fino in fondo ad impegnarci per una politica

infatti, dall'acciaieria di Borgo Valsugana è stata emessa una quantità di diossina 500 volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. Dopo trent'anni di sopportazione e di copertura da parte della Provincia autonomia di Trento, la gente ha detto basta. Ieri sera in una tumultuosa assemblea sono stati resi noti i risultati di un'inchiesta sconvolgente,

(in Valsugana, Trentino orientale, abitano soltanto 50.000 persone). Questa acciaieria, peraltro, scaricava clandestinamente in montagna, poco lontano, sul monte Zaccon, le proprie scorie. È emersa quindi una discarica abusiva piena di metalli pesanti e ora la magistratura finalmente si è mossa: ha aperto un'inchiesta, ha iscritto nel registro degli indagati 12 persone, le quali quattro sono gli ispettori della Provincia autonoma di Trento, che avrebbero dovuto controllare questa attività e che invece sono risultati complici complici degli inquinatori. Lo hanno dimostrato mesi e mesi di intercettazioni ambientali e, soprattutto, di testimonianze. Ora, a seguito di questa inchiesta, come dicono i giornali, la fabbrica è stata posta sotto sequestro, ma con una formula un po' bizzarra: si continuare a produrre con un custode giudiziario. La gente ieri sera si è ribellata dicendo che se è vero che sono stati rovesciati tali veleni, bisogna che la produzione cessi in maniera totale ed immediata. Sono casi che ci ricordano drammi che speravamo superati dall'esperienza passata. Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento è stato

Sembra che la Giunta provinciale adduca come scusante di una certa titubanza la difesa di 117 posti di lavoro. Signora Presidente, non si barattano posti di lavoro con vite umane!